Onorevoli colleghi, l'11 giugno di venticinque anni fa, moriva a Padova l'onorevole Enrico Berlinguer, segretario nazionale del Partito Comunista Italiano. Nato a Sassari nel 1922, godette negli anni della formazione di un contesto familiare intellettualmente ricco, vivace, al centro di significative relazioni personali e politiche. Iscrittosi nel 1943 al Partito Comunista Italiano, fu presentato a Palmiro Togliatti dal padre Mario, avvocato vicino al Partito d'Azione e vecchio compagno di scuola del leader comunista. L'ottima impressione suscitata nel segretario del partito dalle sue qualità valse al giovane attivista sardo una serie di importanti incarichi organizzativi, nel cruciale periodo tra il 1944 e il 1945. I risultati di quella esperienza segnarono, per Berlinguer, l'avvio di una carriera di dirigente politico: segretario dei Giovani comunisti dopo la Liberazione, membro della direzione del partito nel 1948 (a soli ventisei fu eletto deputato nelle elezioni del 1968, capolista della circoscrizione elettorale di Roma. Nello stesso anno, dopo i fatti di Praga, il Partito Comunista Italiano, nella persona del vice segretario Berlinguer, aveva per la prima volta condannato l'intervento sovietico in Cecoslovacchia e nel 1969, alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti, aveva pubblicamente manifestato il proprio dissenso, rifiutando di firmare la relazione conclusiva. Nel 1972, al termine del XII Congresso, Berlinguer fu chiamato a succedere a Luigi Longo come segretario del partito, sulla base di un programma politico che, sul piano interno, proponeva di riprendere la formula togliattiana della collaborazione fra le grandi forze popolari del Paese (socialisti, comunisti e cattolici) e sul piano internazionale esprimeva un indirizzo di lenta, ma progressiva autonomizzazione dalle direttive del Partito Comunista sovietico, in nome delle insopprimibili differenze fra i partiti che operano in Paesi democratici, come il Partito Comunista Italiano, e le formazioni al potere nei Paesi retti da regimi socialisti. La riflessione sugli eventi cileni del settembre 1973, che mostrarono in modo drammatico i rischi ai quali poteva andare incontro una democrazia dalla base politica e sociale troppo fragile, portò Berlinguer a specificare ulteriormente la sua linea, prefigurando quello che egli definì "un nuovo, grande compromesso storico tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano". Si trattava, di fatto, di una esplicita manifestazione di disponibilità a condividere la responsabilità di governo con il partito della Democrazia Cristiana, in nome di una «solidarietà nazionale» che ponesse le istituzioni in grado di fronteggiare le dure sfide di quegli anni alla democrazia italiana: la crisi economica e il terrorismo. L'iniziativa di Berlinguer, rafforzata dal buon risultato elettorale conseguito dal Partito Comunista Italiano nelle elezioni del 1975 e del 1976, si salderà ad analoghe teorizzazioni sviluppate, in quegli anni, da Aldo Moro, conducendo alla nascita, nel luglio del 1976, del primo Governo di «solidarietà nazionale», che si reggeva sulla «non sfiducia» dei parlamentari del Partito Comunista Italiano. Nello stesso anno, Enrico Berlinguer rendeva definitivo lo strappo con Mosca, affermando, davanti al XXV Congresso del Partito Comunista sovietico, il valore della democrazia e del pluralismo, e riconoscendo, in una storica intervista al «Corriere della Sera», l'importanza dell'appartenenza italiana al Patto Atlantico, a riprova dell'autonomia del suo partito dalle influenze sovietiche. Il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, nel momento in cui si prefigurava una fase di più stretta collaborazione al Governo da parte comunista, segnò il passaggio ad una nuova stagione politica: conclusosi il momento di più acuta emergenza, nel quale il Partito Comunista si segnalò fra i protagonisti della «linea della fermezza», la formazione politica diretta da Enrico Berlinguer tornò fra le forze di opposizione. Negli ultimi anni, dopo la fine dell'esperienza della solidarietà nazionale, Berlinguer moltiplicò le prese di posizione sui grandi temi della politica italiana ed internazionale, in molti casi innovando radicalmente rispetto alla precedente tradizione del suo partito: così avvenne a proposito del disarmo atomico, del valore dell'integrazione europea, del dialogo con il mondo cattolico, del rapporto tra morale e politica. Nel suo ultimo discorso, tenuto durante la campagna elettorale per il primo rinnovo del Parlamento europeo, egli dedicò un passaggio significativo alla libertà e alla democrazia come valori assoluti, per il cui perseguimento il Partito Comunista si batteva non soltanto a beneficio proprio e del campo progressista, ma a beneficio di tutti. Un'affermazione che venticinque anni dopo, in un contesto politico di consolidata alternanza democratica e generale accettazione dei valori liberali, potrebbe apparire quasi scontata, ma che invece racchiude in poche parole tutta l'importanza che una figura come quella di Enrico Berlinguer ebbe per lo sviluppo e il consolidamento della democrazia italiana. Egli, infatti, in un momento storico tra i più difficili della vita della Repubblica, seppe mettere il suo indubbio carisma - fatto di rigore, serietà, capacità di parlare agli uomini ed ascoltare i loro bisogni - al servizio di un progetto politico ben definito. Sulla portata dei risultati conseguiti dalla sua azione politica è ancora aperto il dibattito fra gli storici: quel che è certo è che Berlinguer, pur senza aver mai ricoperto incarichi istituzionali e di Governo, va senza dubbio annoverato tra i politici più rilevanti dell'Italia repubblicana. Il Senato della Repubblica, a venticinque anni dalla tragica e prematura scomparsa, rivolge alla memoria di Enrico Berlinguer l'omaggio del ricordo di un grande e appassionato leader politico. Signor Presidente, colleghi, «un uomo introverso e malinconico, di immacolata onestà e sempre alle prese con una coscienza esigente, solitario, di abitudini spontanee, più turbato che allettato dalla prospettiva del potere, e in perfetta buona fede, di cui ci resta un programma sociale, politico, economico, etico e morale non scritto basilare per il futuro democratico e di progresso del nostro Paese». Con queste parole, Indro Montanelli alcuni anni fa rendeva omaggio ad Enrico Berlinguer. Credo sia questo il modo migliore per ricordare la scomparsa di un uomo a venticinque anni dalla morte, il cui valore individuale è stato riconosciuto anche dai suoi più acerrimi avversari politici. Una commemorazione, dunque, senza alcun intento celebrativo né formale e, men che meno, agiografico. Ci domandiamo oggi quale possa essere l'attualità di Berlinguer a distanza di un quarto di secolo, quando i tempi della politica sembrano oggi consumarsi nel breve volgere di momenti e con un panorama complessivo profondamente mutato. Sono passati 25 anni e sappiamo che è cambiato tutto. Il mondo non è più bipolare. È cambiata l'Europa, che non è più divisa, ed è cambiata l'Italia nei suoi connotati. Eppure, ricordare la figura del grande politico e analizzare il suo lascito all'Italia e alla politica di oggi riteniamo abbia un grande valore. Non possiamo dimenticare, ad esempio, che caratteristica peculiare di Berlinguer, che lo fa associare strettamente ad un altro politico di quella stagione, anch'egli morto tragicamente, seppur per diverse ragioni, Aldo Moro, fu proprio la lungimiranza politica, l'aver cercato di guardare agli interessi generali del Paese, mai schiavi del contingente e del giorno per giorno, ma cercando di immaginare e costruire un'Italia migliore. Enrico Berlinguer è stato sicuramente un dirigente amato, e lo si è visto anche in quelle tragiche giornate di venticinque anni fa, quando un intero Paese raccolse il suo ultimo respiro e sentì il dovere di tributargli onore. Fu importante che anche l'onorevole Almirante andasse a rendere omaggio alla sua salma, accolto dai dirigenti del Partito Comunista, dopo anni di tragica contrapposizione. È senz'altro arduo tentare di ricordare la figura di Berlinguer collocandola oggi nell'attuale contesto politico e istituzionale. Arduo anche perché venticinque anni sono troppi per valutare il peso del suo pensiero e della sua attività in rapporto all'oggi, mentre sono pochi per inserirli in una prospettiva storica che lo collochi tra le grandi figure del nostro passato. È più opportuno sottolineare alcune sue scelte e alcuni aspetti della sua persona che hanno impresso segni profondi non solo nella memoria degli italiani che quelle scelte hanno condiviso, ma anche nel dibattito sulle potenzialità, sui limiti, sulle prospettive della democrazia italiana. Mi piace ricordare, innanzitutto, lo sforzo costante di Enrico Berlinguer nel radicare, guardando agli interessi strettamente nazionali, i temi della politica economica, dei modelli di sviluppo della società, del rafforzamento della democrazia, nonostante la forte tradizione internazionalista del suo partito, il suo richiamo costante ai valori della nostra Costituzione, patto fondativo della Repubblica, alla cui costruzione, il suo partito, il PCI, assieme ad altre forze antifasciste, aveva offerto un contributo fondamentale sia nella lotta di Liberazione che nel processo costituente, a sottolineare ancor più il radicamento del comunismo italiano nei fatti fondativi della Repubblica. Il coraggio politico di Berlinguer, che trovava alimento nella profonda convinzione del radicamento nazionale del proprio partito, lo ha portato a schierarsi su posizioni che sviluppavano coerentemente tale visione: l'accettazione della collocazione atlantica dell'Italia e la piena e convinta adesione alla costruzione europea e soprattutto quelle della linea della fermezza nei confronti del terrorismo. La sua intransigenza nel non trattare con le BR durante il rapimento di Moro, nasceva dalla sua profonda convinzione che lo Stato non poteva che essere difeso applicando le leggi, nella cornice costituzionale. Ogni forma di eversione e di violenza politica, tesa a minare la democrazia, come in quei momenti il terrorismo si prefiggeva di fare con le sue azioni, rappresentava per Enrico Berlinguer un pericolo che correvano le masse popolari che tanto avevano lottato per la conquista della democrazia, unico terreno possibile per conquistare e garantire migliori condizioni di vita e di lavoro. La lezione tuttavia che rimane lucidamente attuale è quella legata alla cosiddetta questione morale. Parlando agli intellettuali, in un convegno dedicato ai temi della cultura, anticipò, sorprendendo molti, uno degli aspetti della crisi dei partiti, che è lungi dall'essere completamente risolta ancor oggi. Per Berlinguer i partiti dovevano lasciare più spazio alle dinamiche della società, evitando di presentarsi come eccessivamente invasivi e pervasivi di tutti i gangli istituzionali e sociali. Dovevano riacquistare la loro capacità di attrazione, di aggregazione delle persone attorno a ideali, abbandonando la deriva, che lucidamente intuiva, e che li avrebbe portati a trasformarsi in macchine di potere e di clientela. In questa critica feroce e che allora appariva a molti sconcertante, c'era tutta la tensione ideale che spingeva verso una possibile autoriforma della politica, nel quadro di una profonda fiducia nel sistema dei partiti intesi come soggetti fondamentali della vita democratica. Berlinguer, nell'ambito della questione morale, concepiva l'austerità non come misura politica contingente, ma come un mezzo per ridiscutere in maniera radicale il modello di sviluppo e di società. Per lui austerità significava rigore (anche personale), serietà, efficienza, buon uso delle risorse, lotta contro lo spreco, lo sperpero, l'individualismo sfrenato. I temi della riflessione berlingueriana, oggi, ci richiamano a questioni che stanno nel nostro dibattito politico, e non mi riferisco solo alla questione morale. Nel 1979, su «Rinascita», Berlinguer affermava che era profondamente convinto che la classe operaia «non è assolutamente disposta ad accettare che i suoi soldi vengano utilizzati per rilanciare i vecchi e tarati meccanismi economici che non hanno prospettiva; ma che essa è pronta a fare la sua parte di impegno materiale e morale per interventi che espandano la base produttiva, trasformino le strutture economiche e sociali, avviando a soluzione, in primo luogo, la questione meridionale». Ma tra le tante citazioni che si potrebbero fare delle sue parole, trovo particolarmente significativa una che abbraccia umanità e politica, cioè quando egli diceva che non esiste un modo di essere dato una volta per tutte, ma «un divenire dell'uomo, un cercare di essere, una capacità di abitare nel tempo e nella propria epoca, e di cambiare tenendo forti e saldi i propri princìpi». Penso sia un'indicazione estremamente preziosa, quella di essere capaci di progredire sempre. Ciò che ho cercato sinteticamente di esporre, rappresenta un grande patrimonio di intuizioni e di scelte coraggiose. E oggi non si tratta di stabilire quante di quelle intuizioni e di quelle scelte fossero allora condivisibili o meno. II punto fondamentale è che esse furono sempre, sempre, per Enrico Berlinguer, il frutto di una concezione alta della politica. E ricordarlo oggi, in quest'Aula, è una lezione per noi tutti. Signor Presidente, colleghi senatori, Enrico Berlinguer fu sicuramente un grande leader popolare, attento osservatore e fine intellettuale. Ebbe, tra gli altri, il merito di spingere il PCI oltre la tradizione comunista e filosovietica grazie ad una visione lungimirante ed europeista. L'aria che respirò fin da bambino fu quella dell'antifascismo democratico e liberale che lo portò, a soli 14 anni, ad assumere atteggiamenti contestatari e ad aderire in forma segreta e clandestina al Partito Comunista Italiano di cui diventò poi uno dei massimi dirigenti. Fondamentale nella sua vita fu l'incontro con Palmiro Togliatti, che lo portò inizialmente a ricoprire cariche a livello locale, per poi arrivare in Parlamento. Nel 1943 Berlinguer si iscrisse al Partito Comunista Italiano e ne organizzò la sezione di Sassari svolgendo un'intensa attività di propaganda che lo rese un osservato speciale della questura; da qui varie vicende che lo videro protagonista di arresti e carcerazioni. Dopo il periodo come vice segretario del PCI in Sardegna, Togliatti lo richiamò a Roma; nel 1949 fu nominato segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana, carica che avrebbe mantenuto sino al 1956. L'anno seguente divenne segretario della Federazione mondiale della gioventù democratica, associazione internazionale di giovani marxisti. Membro della segreteria nazionale già nel 1958, ne divenne vice segretario nel 1969 e segretario nel 1972. Eletto per la prima volta deputato nel 1968, si fece portavoce della corrente progressista e popolare del partito. Nominato nel corso del XII Congresso vice segretario nazionale, guidò nel 1969 una delegazione del partito ai lavori della Conferenza internazionale dei partiti comunisti che In tale occasione, trovandosi in disaccordo con la linea sovietica, fonte massima degli indirizzi dell'Internazionale comunista, la presa di posizione inattesa, quanto «scandalosa», fu memorabile: tenne il discorso più critico in assoluto fra quelli che mai leader comunisti abbiano tenuto a Mosca, rifiutando tassativamente la scomunica dei comunisti cinesi e rinfacciando che l'invasione sovietica della Cecoslovacchia (che definì espressivamente la «tragedia di Praga») aveva solo evidenziato le radicali divergenze affioranti nel movimento comunista su temi fondamentali come la sovranità nazionale, la democrazia socialista e la libertà di cultura. Nel 1970 Berlinguer proclamò un'altrettanto inattesa apertura verso il mondo dell'industria: dichiarando che il PCI guardava con favore ad un nuovo modello di sviluppo, inseriva il partito in un dibattito politico-economico fino ad allora considerato tabù per i comunisti. Nel 1973 avviò un nuovo corso della politica del Partito Comunista Italiano lanciando la formula del compromesso storico. Il punto di partenza del ragionamento di Berlinguer fu rappresentato dalla necessità di impedire il costante pericolo di spaccare in due il Paese. Questa tendenza si era manifestata in Italia a partire dal 1969, quando all'attivismo studentesco e operaio si contrapposero la strategia della tensione e il conseguente deterioramento della situazione economica. Le forze reazionarie stavano cercando anche in Italia di creare un clima di esasperata tensione che aprisse la strada ad un governo autoritario o, perlomeno, ad una svolta durevole a destra. Fondamentale fu la sua visione del socialismo democratico che lo portò a contestare apertamente la repressione da parte dell'Unione Sovietica della Primavera di Praga. Altrettanto netta fu la posizione di Berlinguer nel caso dell'ingerenza di Mosca nei confronti dell'Afghanistan e della Polonia. Altro tema cardine della politica di Berlinguer fu la questione morale, ossia la denuncia della corruzione e dello strapotere del sistema dei partiti.

Un tema in cui Berlinguer fu precursore fu quello del decentramento politico, amministrativo e fiscale nel quadro di una maggiore responsabilizzazione dei centri di spesa locale. Nel novembre 1980 lanciò la proposta del Governo delle sinistre, aperto ai laici e ai cattolici progressisti, ma i rapporti con il Partito Socialista andarono sempre più deteriorandosi. Per tutti, infine, deve rimanere il ricordo di un uomo che ebbe indiscussi esempi di lungimiranza politica e seppe arrivare a capire prima fenomeni e questioni che altri intuirono troppo tardi o mai. A quel viso di uomo serio, impegnato, spesso con la sigaretta in mano, un modello comunque, va oggi il nostro più sentito ricordo.

Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, tra le figure di prima grandezza della politica italiana repubblicana Berlinguer rappresenta un caso speciale: lo si potrebbe immaginare oscillante tra momenti di esitazione e di critica e momenti di grande capacità di decisione e di impulso. Sono passati 25 anni dalla sua morte e la sua figura è così complessa, sfaccettata e ricca di implicazioni che la storiografia politica non è ancora stata capace di tracciare una raffigurazione completa. Sono stati scritti molti libri su di lui, sono tematici e riferiti a punti cardine della sua politica (l'atteggiamento di fronte al fattore «K», la questione del compromesso storico, la rigenerazione della politica, la questione morale, l'atteggiamento nei confronti del terrorismo), ma il personaggio ha attraversato così tanti decenni e ha dovuto affrontare così tante questioni, facendolo sempre con un suo stile problematico, che ancora non abbiamo un ritratto, che forse solo la storiografia successiva potrà fare. Non è compito di un intervento in Senato quello di ricomporre il caleidoscopio complesso di tante immagini. Penso che sia più giusto affidarsi alla forte funzione simbolica che quest'uomo

temeva la vittoria di un'opinione pubblica italiana attardata in una visione ottocentesca. La cautela di dirigente politico lo trattenne a lungo; poi, a un certo punto, presa la decisione, si batté con grande energia e la cosa più curiosa è che fu sorpreso dal successo del *referendum*. Trovo in questa sorpresa il segno del carattere dell'uomo che sviluppò a quel riguardo anche una visione autocritica: scoprì e dette, da allora in poi, al protagonismo femminile un rilievo notevole. Scoprì che la società italiana era più matura di quello che avevo temuto. Credo che sia giusto ricordare nei personaggi della politica italiana più i momenti dell'incertezza che quelli della certezza perché questa, dopo tutto, è facile.

anche nei confronti del fattore «K». Alcuni storiografi - di tante scuole, anche del suo orientamento politico - gli hanno rimproverato lunghe esitazioni; altri hanno pensato che invece sia stato troppo coraggioso e troppo impetuoso. Resta comunque il fatto che Berlinguer fu la persona la persona che più di tutte seppe additare una visione critica dei Paesi del socialismo reale e fu tra i più fermi nel momento in cui bisognava avere un atteggiamento di critica di critica serrata degli aspetti degenerativi, chiusi, totalitari dei Paesi dell'Est. La questione del compromesso storico nacque da un accadimento occasionale che poteva non esserci, ma - ahimè! - ci fu, il colpo di Stato in Cile, che ci ricorda che anche la politica internazionale americana non è indenne da critiche. Di fronte a questo evento, Berlinguer colse l'occasione per introdurre un elemento che

tutto sommato, consociativa, ma non credo che quella fosse la critica giusta. Lo ha riconosciuto anche Ginsborg, che, nel suo libro sulla storia italiana, dopo aver criticato la visione del compromesso storico, alcuni documenti che inequivocabilmente mostrano come il senso di allarme di un uomo politico addentro alla scena dovesse essere più forte di quello di chi stava fuori. 12 milioni di dollari ricevuti dall'ambasciatore Graham Martin per influire sulla politica italiana è venuta fuori dopo, ma Berlinguer sicuramente lo sapeva e questo forse giustifica anche un atteggiamento di cautela.

cui cominciò a parlare di capacità di rigenerazione e di rinnovamento della politica di fronte al degradare di quella che lui chiamò per primo questione morale. Non mi attardo su tale argomento perché sono fatti più recenti ma voglio ricordare la persona che, nei confronti della questione morale, era il testimone più indiscutibile. Su di lui non si potevano appuntare critiche personali. Era una persona sobria e disinteressata, tanto che - lo ricordo e forse non tutti lo sanno - non ebbe mai nemmeno l'idea di comprarsi una casa. Ecco, in una situazione di ulteriore degenerazione di taluni aspetti della democrazia italiana, in una condizione in cui ci si avvia - io temo, ma spero che non sia vero - ad un'accettazione sempre più rassegnata di una Repubblica fondata sul conflitto di interessi, Berlinguer rappresenta non solo un uomo privo di conflitti di interessi, ma forse anche privo dell'interesse personale. L'uomo politico capace di incarnare veramente, e con una convinzione che gli è stata riconosciuta intatta, la rappresentanza del popolo senza il vincolo di un interesse personale.

indubbiamente per l'autonomia di pensiero mista ad una certa dose di coraggio, per quei tempi, che ne caratterizzò l'azione politica. Introverso, per certi aspetti quasi duro, Berlinguer ha dato ai comunisti italiani l'impronta europea che questo partito partito cercava di avere già dopo il 1948, quando il cosiddetto blocco popolare, di cui il Partito Comunista era portatore, fu superato dalla coalizione democristiana e repubblicana. Berlinguer è stato un politico di razza, un uomo che ha avuto l'omaggio di un avversario politico come Giorgio Almirante, che guidava un partito fuori dal famoso arco costituzionale. Il leader del Partito Comunista, specialmente dopo il 1974, con il massimo storico per Botteghe Oscure, non osò mai barattare la libertà del suo pensiero e dei comunisti di allora per questioni di mero poltronificio. Conscio del grande risultato, continuò a perseguire quella politica di vicinanza verso il suo popolo, dalle borgate romane alle fabbriche del Nord, ma contestualmente isolando i fanatici che volevano rivoltare lo Stato e che poi si coagularono intorno al terrorismo rosso. Guido Rossa, berlingueriano della prima ora, ne pagò le conseguenze, ma Berlinguer non arretrò di un millimetro, dimostrando altrettanta autonomia di giudizio quando, nel settembre 1977, nel pieno degli scontri di Bologna, arrivò ad accusare gli autonomi e parte dei movimenti giovanili di essere lucidi organizzatori di un nuovo squadrismo, non definibili con altro termine se non quello di nuovi fascisti. Negli anni Settanta Berlinguer proclamò un'altrettanto inattesa apertura verso il mondo dell'industria, dichiarando che il Partito Comunista guardava con favore ad un nuovo modello di sviluppo, introducendo il partito in un dibattito politico economico fino ad allora considerato tabù per i per i comunisti, nella convinzione della necessità di rappresentare un nuovo comunismo, indipendente dall'Unione Sovietica, chiamato eurocomunismo, che si accompagnava alla ferma condanna del Partito Comunista per ogni tipo di interferenza sovietica sia verso l'Italia, che verso altri Paesi, arrivando a dichiarare, attraverso un'intervista rilasciata a Giampaolo Pansa per il «Corriere della Sera», di sentirsi più tranquillo sotto l'ombrello della NATO, anche se non arrivò mai, forse volendolo, ad affrancarsi dai finanziamenti di madre Russia. Berlinguer, forse cercando di dissipare le paure dei cattolici italiani, affermava di voler realizzare una società che senza essere cristiana, cioè legata integralisticamente ad un dato ideologico, si organizzi in maniera tale da essere sempre più aperta e accogliente verso i valori cristiani. La sua sensibilità politica lo portò a considerare, in anticipo sui tempi a venire di Tangentopoli, il tarlo istituzionale della cosiddetta questione morale e, come profondo conoscitore protagonista della storia politica italiana, andava dicendo: «La questione morale esiste da tempo, ma ormai essa è diventata la questione politica prima ed essenziale, perché dalla sua soluzione dipende la ripresa di fiducia nelle istituzioni, la effettiva governabilità del Paese

è stato affidato alle sue ultime parole, pronunciate prima di morire con voce fioca: «Compagni, proseguite il vostro lavoro casa per casa, strada per strada, azienda per azienda». Oggi i *mass-media*, le nuove regole dettate dei vari guru della comunicazione politica, ci insegnano che per esistere politicamente bisogna apparire in perché con il minimo sforzo si raggiungono grandi platee. Ma forse il testamento politico di Enrico Berlinguer si condensa nella frase prima citata, che riporta a serate insonni a discutere di politica in stanze riempite di fumo di sigarette, a comizi nelle piazze nella calura estiva, al rombo dei motori delle macchine che ti conducono di città in città e di paese in paese. Tutto questo, noi della Lega lo facciamo ancora e i risultati si vedono. Evidentemente, Berlinguer aveva ragione.

erano gli anni intorno al '68). Scesi in piazza per la prima volta insieme ai Giovani comunisti, in occasione dell'ingresso dei carri armati sovietici a Praga e del tragico suicidio del giovane Palach.

rincorsa all'aggressione verbale nei confronti dell'avversario politico rischiamo davvero di perdere i contorni dell'identità di ciò di cui stiamo parlando: quelli erano i Giovani comunisti. Il modo con cui il Presidente e i colleghi hanno ripercorso la biografia politica di Enrico Berlinguer ci dà il senso di quanto, pur essendo pienamente uomo del proprio tempo e dunque capace di arrivare fino ad un limite, che era quello di appartenere a quel tempo, quel limite Enrico Berlinguer lo raggiunse dopo un percorso che certamente e straordinariamente innovò nella tradizione del Partito Comunista Italiano, nella storia repubblicana, nella difesa della democrazia italiana. Ed è bene ricordarlo per evitare ancora fraintendimenti nell'uso della parola «comunista» con riguardo all'esperienza del Partito Comunista Italiano, che io trovo improprio: direi assolutamente sbagliato e falso. io non sono qui per ripercorrere solo una biografia, ma anche per ricordare una personalità politica, con un percorso politico difficile e complesso, cui accennava poc'anzi il collega Pardi, che ringrazio. Ho pensato che forse

vivono nella società italiana. Lo voglio fare in omaggio a quella convinzione profonda - ne parlavamo poc'anzi con Vincenzo Vita - propria di Enrico Berlinguer, scienziato della politica, pienamente pienamente consapevole e convinto che la politica fosse una scienza umana. Il riferimento che poc'anzi il senatore Pardi faceva alla sua sorpresa di fronte al risultato del *referendum* sul divorzio

e del riconoscimento che a quel punto andava attribuito alle donne italiane che, soprattutto nel Sud, è bene ricordarlo, avevano mostrato di essere assai più lungimiranti di quanto non fosse stato il crisma di una campagna politica del tutto divisoria ed astratta. L'esperienza di vita concreta delle donne italiane aveva condotto ad un risultato di cui per primo Enrico Berlinguer si stupiva, salvo poi valutarne il peso ed elevarlo quindi a valore della propria azione politica. Voglio poi parlare di un aspetto tipico di chi considera la politica una scienza umana e che trascende l'idea, propria di Berlinguer ma direi propria del Partito Comunista Italiano, che i partiti avessero anche una funzione pedagogica, non soltanto l'intellettuale collettivo, espressione di cui abbiamo tante volte letto e che pure fu capace di di creare una trama molto fitta nei confronti di un fenomeno emergente come il terrorismo. Enrico Berlinguer credeva che il partito potesse essere creatore di una consapevolezza e di e di una conoscenza collettive, capaci di fronteggiare anche i grandi eventi e le questioni che attraversavano, questa volta tragicamente, la storia d'Italia.

impersonato dai nostri padri e dalle nostre madri (mio padre era proprio coetaneo di Berlinguer) agitava non soltanto le discussioni familiari, ma anche il nostro animo, l'animo di quei ragazzi, e forse ancor di più di quelle ragazze, che non si riconoscevano nei modelli e nel modo con cui la vita era stata impostata. Avvertivamo con fastidio, talvolta proprio con viva insofferenza, i modelli educativi che i genitori, sulla base della propria esperienza di vita, tentavano,

qualcuno la Resistenza e la gioia della Repubblica e della democrazia. Bene, lo strappo, come viene definito, questo valore assoluto della democrazia e dei valori repubblicani, questa rivendicazione del catalogo dei diritti delle libertà come bene supremo era un terreno di incontro tra la generazione di mio padre e la mia generazione per il tramite della lezione di Berlinguer. Allo stesso modo, la lezione dell'austerità, della sobrietà e del rigore per noi che avevamo genitori (e li abbiamo ancora, qualcuno di noi) che venivano dalla guerra e che del rigore, della sobrietà e dell'austerità avevano fatto un parametro identitario dell'educazione,

vita individuale, era un modo per comprendere il valore di quella educazione e per non avvertirla come straniante ed estranea rispetto alla nostra esperienza di vita.

le figure delle nostre madri ci apparivano talvolta scolorite, sottomesse, non pienamente consapevoli di sé e del proprio valore. Enrico Berlinguer

essere capaci di interpretare la politica come qualcosa che non è figlia di una strategia o di un tatticismo, che non guarda all'interesse personale (lo diceva poc'anzi il senatore Pardi, ma questo secondo me va da sé),

dovrebbe comunemente fare e troppo spesso, me lo si lasci dire, non è proprio capace di fare. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Popolo della Libertà si associa al ricordo commosso della figura di Enrico Berlinguer. Queste occasioni tendono giustamente e doverosamente a mettere in luce i lati positivi dei protagonisti e delle personalità che hanno contrassegnato la nostra storia repubblicana. L'intervento della collega Finocchiaro non poteva non essere caratterizzato anche da accenti personali, familiari e generazionali: lo comprendo perfettamente e mi sarei trovato nella stessa condizione umana e psicologica se avessi dovuto commemorare figure come Giorgio Almirante o altri leader che, per la mia esperienza personale e per la mia generazione, possono rappresentare quello che Enrico Berlinguer ha rappresentato per la sinistra e per le generazioni che si sono formate sotto quella guida. In questi giorni numerose sono state le occasioni di ricordo di Berlinguer e sono state promosse in vari ambiti, con protagonisti di diverse provenienze. Ha suscitato attenzione il fatto che personalità che hanno vissuto a destra hanno avuto espressioni di grande considerazione. Nei giorni scorsi è stato Gianfranco Fini - che oggi è Presidente della Camera, ma che ha

pagine importanti di quella esperienza: gli strappi, le critiche a Mosca e anche quell'affermazione, che ha avuto una grande rilevanza nel dibattito politico italiano, che Berlinguer fece nel 1981, quando dichiarò che si era esaurita la spinta propulsiva della Rivoluzione di ottobre. C'è voluto del tempo perché il dibattito a sinistra proseguisse. Eravamo nel 1981, quindi ben prima della caduta del muro di Berlino, che avvenne otto anni dopo; Berlinguer, scomparso nel 1984, non ebbe la possibilità, per un destino così tragico, di confrontarsi con quegli eventi. Tuttavia, il pronunciamento del 1981 rientrava

Schifani, aprendo i nostri lavori, ha sottolineato con solennità il ruolo e l'importanza della figura di Berlinguer. In questi giorni, paradossalmente come sempre accade, altri hanno dato letture diverse. Mi ha colpito, nei giorni scorsi, un articolo di Giampaolo Pansa, giornalista e storico che ebbe frequentazioni giornalistiche e interviste con Berlinguer, che invece ha usato accenti un po' più critici e severi. Ricordiamo tutti le pagine della lotta al terrorismo. Credo che verrei meno alla sincerità di un'occasione di ricordo, che deve essere formale, solenne e rispettosa, se non ricordassi anche altre pagine che restano scritte nella storia italiana. Era il 1975 quando Enrico Berlinguer ancora ricordava che «nei Paesi socialisti si registrano ulteriori miglioramenti del tenore di vita dei popoli e nel loro sviluppo civile e culturale. In quei Paesi», diceva Berlinguer, «esiste un clima morale superiore». affermazioni che forse nel 1981 Berlinguer non avrebbe fatto e che la sinistra di cui egli era stato il capo in gran parte non ha fatto; altri hanno continuato a pensarla così. Anche la vicenda del terrorismo ebbe uno spartiacque drammatico e lacerante nel sequestro Moro, nel 1978, quando un intero arco politico si schierò con coraggio e sofferenza contro ogni trattativa e cedimento e Berlinguer, facendosi carico, come Cossiga e altri, di quel dramma, tenne quella posizione. Negli anni precedenti troppe volte la sinistra era stata incerta di fronte all'irrompere delle Brigate Rosse. Ricordiamo ancora i titoli sulle sedicenti Brigate Rosse e una discussione che anche il partito di Berlinguer dovette maturare a lungo, proprio con il sequestro Moro, prima di assumere una decisione di netta condanna. Ricordo i titoli e le ambiguità degli anni precedenti e non posso non riferirne anche in questa occasione. Quando si parla di Berlinguer giustamente si ricordano anche i richiami alla questione morale. Personalmente ho sempre avuto un grande rispetto della figura del militante: un leader politico che cade durante una manifestazione politica, come accadde a

vicenda drammatica, accresciuto il rispetto non solo da parte di coloro che avevano le sue stesse idee, ma da parte di tutti gli italiani e, certamente, da parte di chi appartiene ad una comunità politica e quindi, più di altri, si immedesima nello sforzo quotidiano, spesso non compreso da molti cittadini, della militanza, dell'andare in giro e del predicare le proprie idee, quali che siano. Ebbene, rispetto alla questione morale, tutti ricordiamo i richiami di Berlinguer e sono il primo a dire che sotto il profilo personale gli insegnamenti che Berlinguer ha trasmesso al suo partito ed anche la sua famiglia sono stati indubitabili: rigore, l'onestà personale nessuno li ha mai messi in discussione. Forse, talvolta a sinistra si è sottovalutato un confronto sulla questione morale che avrebbe dovuto ricomprendere anche altre vicende. Conosciamo molte questioni esplose con Tangentopoli, ma gli intrecci tra il Partito Comunista dell'epoca, diretto da Berlinguer, i finanziamenti che provenivano da Mosca, gli intrecci con alcune organizzazioni cooperativistiche hanno determinato un flusso di finanziamenti illeciti di quel partito - anche sotto la guida di Berlinguer - che noi non possiamo dimenticare.

«Occorre ammettere che ci distinguiamo dagli altri non perché non siamo ricorsi a finanziamenti deprecabili, ma perché nel ricorrervi il disinteresse personale dei nostri compagni è stato assoluto». che ogni tanto andrebbe riletto, compare anche questa affermazione e se noi la cancellassimo non daremmo onore alla verità della storia, in cui c'è certamente l'omaggio al militante, il rispetto ad un protagonista della vita politica italiana. Ciò però non può farci dimenticare il dibattito delle idee, idee anche confutabili, discutibili (non voglio dire errate) che furono interpretate e divulgate. Anche sotto il profilo della questione morale dobbiamo distinguere l'onestà individuale dei comportamenti da un sistema di finanziamenti illegali che riguardò anche il il Partito Comunista diretto da Enrico Berlinguer. Non faremmo un omaggio serio e sincero se ci limitassimo agli aspetti agiografici. La storia italiana è piena di luci e di ombre. L'epilogo di Berlinguer rappresenta certamente una pagina che tutti ricordiamo con commozione e con

a chi, non essendo sufficientemente informato, pensasse che oggi occupandoci dell'argomento contabilità di Stato, ovvero di una riforma della stessa,

disposte ed approvate dal Parlamento italiano allorché nacque lo Stato italiano, a firma del deputato Cambray-Digny riguarda l'impalcatura e la costruzione della Ragioneria dello Stato. Il che significa che non c'è Stato se se non c'è un valido apparato contabile di rilevazione e di esposizione dei dati

Lo Stato di diritto che allora non c'era oggi la fa da padrone. La pressione fiscale che evidentemente è lievitata, così come era d'obbligo, con la nascita e la dilatazione dello Stato sociale ha fatto sì che notevoli fossero le risorse dello Stato destinate al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Di qui la necessità di una sempre maggiore vigilanza, di una sempre maggiore rendicontazione, di una migliore rendicontazione che riferisse dei piani, dei progetti, dei programmi, del loro divenire, della efficacia, efficienza ed economicità, così come si usa dire oggi. adeguamento dell'apparato contabile in funzione dei cambiamenti istituzionali e delle condizioni dei conti pubblici che, per fatti che oggi non è opportuno rilevare, hanno subito un appesantimento che non ha eguali nella storia d'Italia. Bilancio che non fosse articolato per capitoli, articoli e lettere, così come per le poche risorse allora era necessario fare, ma che esponesse anche le missioni, i programmi, la spesa e il risultato delle stesse. Bilancio che non fosse solo del nucleo centrale che allora era solo e solitario, ma che fosse anche di tutti i rami della pubblica amministrazione, di tutti quelli che genericamente vengono denominati centri di spesa, che sono tanti e che a momenti si è avuto la sensazione fosse impossibile controllare e fotografare. La necessità di contenere il disavanzo pubblico e quindi stagnare il divenire della pressione fiscale, che ha raggiunto quello che De Viti De Marco chiamava il «punto di rottura» al di là del quale o si fugge necessariamente l'obbligo fiscale e si va verso l'evasione oppure ci si astiene dal lavoro. Bilancio annuale e pluriennale perché la velocità del divenire della spesa è tale che un arco temporale di un anno non è sufficiente a dare contezza del suo divenire e della sua utilità.

poi favorevoli anche al controllo rigoroso da parte del Parlamento e all'impegno del Governo per un comportamento elastico, come si addice ad una grande spesa, non scordarsi mai che la Ragioneria generale dello Stato fu sempre, è e deve rimanere la vestale del bilancio pubblico. Essa non è del Governo ma dello Stato,

conto della serva, risulta evidente che per far arrivare il nostro debito pubblico alla media europea in rapporto al PIL, avremmo bisogno di una finanziaria moltiplicata per sei, dunque sei finanziarie normali, per il prossimo mezzo secolo. È evidente a tutti che si tratta di un'operazione assolutamente impossibile.

per i parlamentari e per gli uffici dei dati in formato telematico. Sembra una cosa assurda, ma ad oggi non abbiamo la disponibilità di un *file* di Excel con i dati del bilancio dello Stato; sembra davvero una barzelletta, ma così è. Ebbene, senza avere la contezza e senza avere i dati elaborabili, è chiaramente impossibile fare una valutazione attenta di come vengono spesi i soldi dei contribuenti. Quindi già questo è un enorme passo avanti. Il lavoro però non finisce qui: il provvedimento, dopo aver passato il vaglio del Senato, passerà alla Camera dei deputati dove sicuramente ci saranno ulteriori modifiche; penso in particolare al sistema della Tesoreria, che ci pare un po' troppo pesante e centralizzato, anche e soprattutto nell'ottica della riforma del federalismo fiscale, però avremo modo di approfondire ulteriormente questi temi. Comunque è assolutamente apprezzabile il lavoro di concerto operato in Commissione e tra i colleghi, che ha portato all'elaborazione di un testo condiviso e che sicuramente è un'ottima base di partenza.

ci troviamo ad esaminare un provvedimento complesso per l'ampiezza delle tematiche affrontate e la specializzazione dei contenuti estremamente tecnici, che affiancano ed incidono in maniera rilevante su questioni più squisitamente politiche ed istituzionali, come, ad esempio, il Parlamento come legislatore e controllore, il *continuum* maggioranza-Governo, il vincolo costituzionale di copertura dei nuovi o maggiori oneri. Un testo che già nella versione originaria era strutturato per essere una riforma, un'altra importante riforma promossa e realizzata da questa maggioranza. Il testo presentato in Senato, infatti, già conteneva adeguate risposte alle questioni critiche - che a volte per chiarezza sarebbe meglio indicare come carenze vere e proprie - evidenziate, ovviamente non solo negli ultimi tempi, dalla delicata situazione dei conti pubblici, dall'evoluzione dell'assetto istituzionale, dalla declinazione della cultura del risultato e della responsabilizzazione nella pubblica amministrazione e, non da ultimo, dalla trentennale applicazione della disciplina contabile stessa. Basti pensare, ad esempio, alle norme per un governo unitario della finanza pubblica, a quelle che modificheranno le prossime sessioni di bilancio, mutuate in parte dalla recente legge finanziaria 2009 che ha già evitato quella balcanizzazione del bilancio dello Stato, come ebbe a dire il senatore Pichetto Fratin, relatore di quel provvedimento. Un testo che la Commissione ha ulteriormente migliorato, devo dire anche con la partecipazione responsabile e fattiva dell'opposizione, pur con ruoli ed espressioni differenti. Ma va certamente ascritto a questa maggioranza il merito di aver creduto, voluto, ricercato questa riforma per il bene del Paese; una riforma che da trent'anni attendeva di essere realizzata e che questa maggioranza riuscirà a condurre in porto. Il lavoro della Commissione si è fondato sulle interessanti audizioni di rappresentati delle istituzioni e del mondo accademico, che hanno messo a fuoco e fatto risaltare gli aspetti critici, metodologici ed operativi che hanno caratterizzano l'attuazione della disciplina contabile in vigore. Pertanto, non posso che esprimere un forte apprezzamento per le soluzioni cui è pervenuta la Commissione, convinta delle efficaci innovazioni apportate al trentennale impianto vigente, il grande lavoro del presidente Azzollini, che ha potuto condurre questo dibattito accurato, approfondito e proficuo. Tuttavia, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni su qualche aspetto attinente la legge di bilancio, che mi sembra sia rimasto un po' sospeso. Non intendono essere delle spiegazioni, ma più problematicamente spunti di riflessione, considerazioni personali che forse vale la pena approfondire, sottoporre ad un supplemento di indagine da parte di questa Assemblea, e magari anche della Camera dei deputati nel prosieguo dei lavori parlamentari. Alcune questioni che incidono su rilevanti aspetti politici, sulle regole, scritte e non scritte, per la decisione più importante di politica economica, da costruire nelle istituzioni competenti e tra di esse. La prima di tali questioni attiene alle possibili ricadute del nuovo ruolo assunto dalla legge di bilancio. Già nel corso dell'ultima sessione di bilancio, il disegno dì legge di bilancio è stato oggetto di una rinnovata attenzione, perché ha assunto un ruolo differente nell'ambito della manovra finanziaria ed instaurato un diverso rapporto con l'altro strumento della manovra, la legge finanziaria, da adesso legge di stabilità. Il disegno di legge di bilancio, invece, è divenuto lo strumento con il quale, in una fase successiva al richiamato decreto-legge n. il Governo ha definito e sottoposto alla valutazione del Parlamento le scelte allocative della spesa, utilizzando l'impianto classificatorio introdotto l'anno precedente, le nuove missioni, i nuovi programmi. Uno strumento, inoltre, flessibile, che consente cioè alle amministrazioni di rimodulare, pur con alcuni limiti, le dotazioni tra i programmi di ciascuna missione. Rimodulazione possibile, ricorrendo anche alla modifica delle autorizzazioni di spesa ad esse sottostanti, indicando di quali autorizzazioni si tratta e il corrispondente La riconsiderazione del bilancio come strumento di politica finanziaria porta ad interrogarsi sulla opportunità di estendere il limite della compensatività delle variazioni eventualmente apportate. Ora, infatti, le variazioni compensative delle eventuali modifiche possono essere effettuate entro l'aggregato missione, ma non sarebbe più logico estendere l'ambito di compensatività tra le risorse a tutto lo stato di previsione di quel Ministero, ovvero spostarlo ancora più in avanti a tutto il bilancio? Inoltre, dato il mutato rapporto con la legge finanziaria non sarebbe più congruo trasportare da quest'ultima le tabelle, al fine di raggruppare nel disegno di legge di bilancio tutte le decisioni che hanno a che fare con i numeri, con gli aspetti quantitativi delle norme di spesa? Un altro aspetto su cui vorrei esprimere qualche considerazione è la presenza nella pubblica amministrazione di differenti metodologie e criteri contabili, molteplicità che ha imposto la ricerca di una necessaria armonizzazione, che si traduce poi nella trasparenza, omogeneità e coerenza dei dati di bilancio. Così il provvedimento prevede in due diversi articoli - per i quali si auspica un necessario raccordo una delega al Governo per affiancare alla contabilità finanziaria, ai fini conoscitivi e in via sperimentale, un sistema di contabilità economico patrimoniale, funzionale alla verifica dei risultati. Ha un senso, però, in una riforma così ambiziosa, riproporre una situazione di compresenza di sistemi contabili diversi, seppure in via sperimentale ed a fini conoscitivi? La compresenza è sembrata - anche a qualche autorevole personaggio sentito in Commissione - più spesso non completamente soddisfacente Ma allora quale strumento utilizzare? Ce ne è uno buono per tutte le esigenze? Probabilmente no. In questa fase, allora, non dovremmo forse ragionare sull'obiettivo o sugli obiettivi che intendiamo raggiungere, riflettere sui vantaggi e gli svantaggi delle diverse logiche contabili e scegliere, in via definitiva, uno strumento, quello più adeguato allo scopo? Da ultimo, se le rappresentazioni contabili hanno diverse finalità e dipendono dal fenomeno che si vuole rappresentare, perché non pensare alla possibilità di affrontare, anche nel prosieguo, ulteriori tipologie di bilancio e di sistemi contabili? Penso ad esempio al bilancio del cittadino, che è utente e contribuente, elettore e controllore delle politiche pubbliche. Articolato per portatori d'interessi e interlocutori sociali, diverso dal bilancio sociale, potrebbe essere uno strumento di trasparenza, conoscenza, divulgazione e coinvolgimento di chi, forse anche con sacrificio anzi senza dubbio - paga le tasse e ha il diritto di comprendere per poter valutare e giudicare come vengono utilizzati i suoi soldi. In questa logica, peraltro, potrebbe trovare spazio anche un altro strumento contabile interessante, quello del bilancio territoriale, volto a dare contezza delle risorse pubbliche impiegate in quella specifica area, per poter misurare e apprezzare i flussi di spesa correlati al carico fiscale e tributario, nonché i risultati reali conseguiti in termini di effetti e di impatto sulla spesa e soprattutto a quella creazione di valore che è un altro degli obiettivi delle politiche di bilancio. Potrebbe essere, ad esempio, uno strumento esempio, uno strumento urgente da adottare nelle aree metropolitane, Comuni o Province che siano. Si tratta in fondo di ragionare su come valutare l'incremento nella creazione del valore economico e sociale, che riempirebbe di ulteriori contenuti il federalismo fiscale e finanziario rendendolo ancora di più una grande riforma: quella alla quale puntiamo con grande convinzione. Come ho detto, mi sembra che valga approfondire questi aspetti, senza posizioni preconcette e, soprattutto, evitando di inseguire il mito della riforma perfetta. Troppo spesso, infatti, sono state attuate regole e strumenti che introducevano a cambiamenti, ma ciò non ha significato cambiare automaticamente i comportamenti, in questo caso delle pubbliche amministrazioni nelle loro modalità gestionali. Se le regole non entrano nella vita delle persone, se non si incarnano nella vita del Paese e nella sua identità, restano scritte sulla carta, come tante altre volte è accaduto, e piano piano sfumano, non vivono e si perdono, e perde soprattutto il buon legislatore. Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice Ministro, è stato già detto molto nel dibattito che si è svolto sia in Commissione che in Aula sulle ragioni che hanno determinato l'esigenza di pervenire a questa riforma e sulla portata innovatrice della stessa.

un'esigenza, quella appunto di riformare la legge di contabilità, che è andata vieppiù maturando sulla base di dati di fatto che sono largamente condivisi e che sono rinvenibili nella crescente ipertrofia della legge finanziaria, così come si è articolata nel corso degli anni, nella scarsa capacità della legge stessa di incidere sui macroaggregati della finanza pubblica, concentrandosi, invece, sugli effetti marginali recati dagli interventi delle varie leggi finanziarie, nel progressivo scadimento della qualità

pure in condizioni molto difficili, si evitò il ricorso alla fiducia. Inoltre, il complesso di problemi che è andato manifestandosi nel corso degli anni ha prodotto una sostanziale modificazione dell'ordinato svolgimento del processo legislativo e anche dell'organizzazione dell'attività del Parlamento nel suo complesso: la lentezza dell'*iter* di approvazione delle leggi, le contraddizioni interne alle varie maggioranze hanno portato negli anni alla sostanziale modificazione dell'assetto costituzionale nel processo

ai decreti-legge e ai voti di fiducia, dall'altro, le finanziarie *omnibus* quale strumento di concentrazione della volontà legislativa e talvolta anche di compensazione tra le diverse istanze interne alle varie maggioranze. Gli effetti che sono stati registrati sui conti pubblici sono stati virtuosi quando al centro della legge finanziaria e della legge di bilancio è stata posta la missione della correzione dei saldi e del risanamento. Sono state ricordate le leggi del 1992 e del 1996,

Il bilancio veniva considerato uno strumento di registrazione dei tendenziali a legislazione vigente ed era sostanzialmente marginalizzato quanto l'attenzione alla capacità di incidere sull'andamento dei conti

riforma che viene recepita in modo organico da questo testo normativo; poi, conseguentemente, è stata riservata maggiore attenzione allo strumento del bilancio rispetto alla legge finanziaria.

di bilancio, così come si era determinata nel corso degli anni. Nel riformulare la struttura del bilancio nei termini che ho illustrato e nell'avviare quest'opera di revisione ci si avvide che era l'intera sessione di bilancio

in larga parte peraltro contenuti in questo provvedimento legislativo, nell'intento di passare poi alla stesura di un testo normativo Si trattava, in sostanza, di tradurre in norma un progetto che era già compiuto, un impianto già definito. Ricordo il contributo che a quel dibattito diedero il presidente Azzollini ed il vice ministro Vegas, all'epoca componenti della Commissione bilancio. In quelle condizioni, politiche e numeriche, e stante anche la natura del provvedimento - si tratta, come ci è ampiamente noto, di regole istituzionali attuative di principi costituzionali che devono durare nel tempo - veniva sollecitato l'apporto ed il consenso dell'allora opposizione, oggi maggioranza. Solo così si poteva procedere alla riforma due anni fa. Oggi, a parti invertite, è avvenuta la stessa cosa. Raccogliendo quelle idee, e quelle dei tecnici e degli studiosi di contabilità pubblica, oggi come allora la maggioranza ha sollecitato un apporto, un consenso dell'opposizione. La posizione delle maggioranze, quella di allora e quella di oggi - diverse, come è noto - non è mutata; l'atteggiamento delle opposizioni, quella di allora e quella di oggi, è mutato.

di concentrarsi sui contenuti di merito con un lavoro molto importante e prezioso, che è stato fatto per larga parte in Commissione e che, per altra parte, verrà compiuto - mi

Anche qui ci sono analogie con il passato. Si tratta di un atteggiamento fatto di confronto, proposte di condivisione, laddove è stato possibile, di votazioni di emendamenti, in Commissione e in Aula, quasi sempre all'unanimità su proposte importanti e condivise, a volte differenziate; ma ciò fa parte della normale dialettica Il voto finale è parametrato all'esito dell'esame nel merito, al contenuto conclusivo del provvedimento. Ciò è avvenuto sul provvedimento per il federalismo fiscale e avverrà, considerando appunto l'esito e il confronto conclusivo in Aula, in Aula, per la riforma della sessione di bilancio e della legge di contabilità. Ho voluto ricordare queste cose, che sono ampiamente note, per dire che la prossima volta che sentiremo dire in questa Aula da esponenti della maggioranza o del Governo che l'opposizione si rifiuta di formulare proposte o si sottrae ad un confronto di merito mi metterò a urlare, perché queste due importantissime riforme (federalismo fiscale e legge di contabilità) sono state fatte con questo metodo. Sicuramente anche grazie alla volontà di confronto e all'apertura del Governo e della maggioranza, ma - mi permetto di aggiungere - soprattutto in virtù di un atteggiamento responsabile di merito ed improntato alla cura degli interessi generali che l'opposizione ha privilegiato e messo in campo. Il resto delle

dal contenuto della legge finanziaria; non sarà possibile, così com'è avvenuto già per il decreto-legge n. 112 del 2008, inserire nella legge di stabilità norme che riguardano lo sviluppo economico. è nota: i problemi che si erano manifestati nel corso degli anni e di cui parlavo all'inizio derivavano dal fatto che attraverso norme relative allo sviluppo economico a volte, in virtù di questa possibilità, si introduceva nella legge finanziaria di tutto, generando quella ipertrofia cui mi riferivo.

nel testo licenziato dalla Commissione: si è deciso di vietarle, a meno che non abbiano rilevanti effetti finanziari diretti che, quindi, ne consentano l'ingresso nella legge di stabilità. Ebbene, io ritengo che si dovrebbe fare un'ulteriore riflessione: perché non consentire l'introduzione, limitata, delle norme per lo sviluppo economico con la stessa impostazione che riguarda le norme ordinamentali ed organizzatorie? Il corollario dell'estromissione dalla legge di stabilità e dalla legge finanziaria delle norme per lo sviluppo doveva essere infatti - e in questo senso si è mossa una nostra precisa proposta - l'indicazione di tempi certi per l'approvazione dei disegni

dei collegati, il che non garantisce che le norme relative allo sviluppo economico, quelle che incidono sui conti pubblici

di inserire nella legge di stabilità norme per lo sviluppo, purché esse siano strettamente collegate all'esigenza di conseguire gli obiettivi conseguire gli obiettivi di finanza pubblica oggetto della legge di bilancio e della legge finanziaria. Vi sarebbe poi da riflettere sul fatto che i collegati, in realtà, così come abbiamo visto nel corso di questi mesi, sono diventati tante piccole (e neanche tanto piccole) finanziarie. ciò che si è deciso di non includere nella legge finanziaria è poi rientrato nei collegati nei modi che sappiamo. Cito per tutti il disegno di legge sullo sviluppo e sul processo civile, che contiene un volume enorme di disposizioni disomogenee tra loro e non tutte esattamente ricollegabili al contenuto della manovra e alla risoluzione di approvazione del DPEF. Ugualmente, cito il disegno di legge sull'energia: in esso c'era di tutto e soltanto la nostra iniziativa, finalizzata ad arginare l'emendabilità di quelle disposizioni di legge sulla base del Regolamento del Senato, ha consentito di contenere, in parte, quella spinta a rigonfiare i testi normativi. In tal modo si è dimostrato che non è sufficiente mutare la struttura della legge finanziaria per arginare la tendenza alle leggi*omnibus* da parte del Parlamento.

modalità di copertura delle leggi, a proposito delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del disegno di legge al nostro esame, in particolare nel comma 10, che prevede

il capitolo di spesa si sia esaurito, scatta, sulla base della previsione legislativa a monte, una clausola di salvaguardia che consenta di integrare la copertura attraverso attraverso le misure contenute nella clausola di salvaguardia stessa. Ho richiamato questo punto per dire che, a mio modo di vedere, dalla corretta applicazione di questa norma, che mi auguro venga ulteriormente dettagliata in fase di decreti delegati, dipende molto del successo della nuova struttura legge di stabilità e della legge di bilancio. È infatti evidente che, nel caso dei diritti soggettivi, l'applicazione tempestiva e rigorosa della norma in esame potrà costituire garanzia dell'equilibrio

una maggiore efficacia della disposizione, prevedendo anche qualche meccanismo automatico di relazione al Parlamento e di introduzione di sanzioni. Farò un esempio attualissimo: che cosa succederà quando i fondi per il terremoto,

Ipotizzando che quella legge andrà in vigore, quando ciò si verificherà - e certamente si verificherà se non vi saranno interventi di integrazione delle risorse finanziarie come funzionerà questa clausola di salvaguardia? Non è il caso di prevedere un obbligo per il Governo di relazionare in ogni caso al Parlamento e di adottare iniziative conseguenti allorquando le risorse stanziate si sono esaurite?

richiamo l'assoluta positività dei meccanismi di controllo e trasparenza tecnici e parlamentari introdotti, e mi auguro che ci sia un buon esercizio della delega attribuita al Governo e, soprattutto, una successiva buona prassi parlamentare, che consenta di applicare le norme e i principi recati in questa legge di riforma. Se funzionerà,

quello che stiamo discutendo oggi in quest'Aula non è un documento tecnico o una legge di contabilità di interesse pressoché esclusivo di alcuni esperti o pseudo tali o di pochi addetti ai lavori: è la vera pietra d'angolo della democrazia e della libertà per tre ragioni molto semplici. luogo, i dati statistici, in particolare quelli che riguardano la finanza pubblica, sono il primo bene pubblico collettivo; luogo perché la certezza dei conti pubblici significa un corretto confronto tra maggioranza e opposizione nel merito dei provvedimenti e non nei giochetti numerici, qualunque sia il ruolo di maggioranza e opposizione che potrà alternarsi nel tempo; il terzo elemento per il quale questa è la pietra d'angolo della democrazia e della libertà è perché nel rapporto tra Stato e cittadino se non vi è certezza di numeri evidentemente non vi è certezza nel rapporto concreto tra ciò che il cittadino paga e ciò che lo Stato, in tutte le sue articolazioni, fornisce come servizio ai cittadini. Per questi motivi sono molto orgoglioso, ancora di più oggi, del mio Governo, del mio partito, che si chiama Popolo della Libertà, perché nel nome del partito è incarnata questa pietra d'angolo. E sono orgoglioso, di fronte a fin troppe anime candide, che questo provvedimento, che incarna tali princìpi, sia fatto da un Governo di centrodestra nel momento in cui è maggioranza politica.

Questo è il merito del Popolo della Libertà, della coalizione di centrodestra e di questo Governo Berlusconi. Parliamoci francamente:

In trent'anni, con l'articolo 81 della Costituzione, con la legge n. 468 del 1978 che vincolava esclusivamente i saldi di bilancio,

nefasto risultato? Prendo atto della correttezza e della disponibilità dell'attuale opposizione, sia in Commissione bilancio sia in Commissione finanze, e probabilmente anche in Aula. Ma va ricordato che questa riforma dovrà impedire ciò che è avvenuto pochi mesi fa nelle Aule parlamentari: cioè che un Governo, falsificando i conti, carichi gli italiani di tre punti di pressione fiscale in più e sperperi quei 50 miliardi di tasse in più in mille rivoli di spesa, lasciando le condizioni dei saldi finanziari peggiori di quando inizialmente aveva avuto il mandato! Questa è la storia-cronaca degli ultimi due anni. Quindi è molto positivo che ci sia questo clima di collaborazione, ma non va taciuto

Cari colleghi, nel corso delle indagini conoscitive svolte ed in corso presso la Commissione finanze, documenti formali della Corte dei conti, audizioni formali del Dipartimento delle politiche fiscali, e di altri settori dell'*Authority* hanno messo per iscritto e sottolineato a voce che nelle attuali condizioni circa 40-45 miliardi di spesa pubblica sono assolutamente aleatori. del Dipartimento delle politiche fiscali ieri nel corso di un'audizione ha detto ed ha precisato il metodo con il quale vengono valutate le previsioni di entrate e non è stato in grado di dire come mai, seguendo quel metodo, nel 2006 si sarebbe ottenuto un certo numero, come mai quel numero uscito dal Dipartimento fiscale è entrato diverso nei documenti ufficiali presentati all'Aula dal precedente Governo. Non lo dico per polemica, ma per sottolineare l'importanza di questa riforma ed il merito del Governo e del centrodestra che assume queste responsabilità quando è al Governo e quando è maggioranza. illustrare alcuni punti, signora Presidente, che nel corso poi della discussione degli emendamenti in Aula potranno essere meglio articolati. la legge n. 468 del 1978 aveva ed ha due difetti sono quelli che hanno consentito il raddoppio del debito pubblico in questi anni. Il primo difetto è che quella legge vincola soltanto i saldi finanziari e lascia libero qualunque Governo di ottenere uno stesso saldo o con più entrate e più spese o con meno spese e meno entrate. È un punto determinante quello dell'equilibrio finanziario, ma non esaurisce la politica economica; anzi, l'equilibrio finanziario è l'inizio, il punto di partenza di una seria politica economica che nelle Aule parlamentari e nel Paese spieghi chiaramente quanto si preleva, quanto si spende, come si preleva e come si spende, a parità di deficit. Allora il primo punto è proprio questo: far chiarezza tra l'andamento tendenziale dell'economia ed il conseguente andamento tendenziale della finanza pubblica;

sia del quadro macroeconomico che della finanza pubblica. Il secondo difetto della legge n. 468 è infatti che non si calcola quale effetto della correzione della finanza pubblica viene a determinarsi sull'andamento economico. Negli anni scorsi abbiamo avuto l'assurdo di documenti, DPEF e relazioni previsionali e programmatiche che indicavano un andamento del prodotto interno lordo tendenziale identico all'andamento del prodotto interno lordo programmatico dopo la manovra di correzione. Che senso ha fare una politica economica che nei dati ufficiali non ha alcun effetto sull'economia? Quindi, signora Presidente, dai saldi occorre passare al totale delle entrate e delle spese, vincolando il Governo ad indicare questi numeri e la pressione fiscale nell'arco di tre o quattro anni.

però un unico punto da chiarire: proprio perché ci stiamo avvicinando alla realizzazione del federalismo fiscale, a maggior ragione il Parlamento deve avere un

dei bilanci pubblici sia assegnata sulla base delle competenze già esistenti ad un'autorità indipendente. Sono due elementi separati: un conto è un Parlamento in grado di fare analisi, un altro è la certificazione dei bilanci di tutto il comparto pubblico. Con la realizzazione del federalismo fiscale, ho paura

di tanti bilanci e di tanti numeri, con una responsabilità assegnata ai singoli Governi ma senza alcuna responsabilità di avere quei dati certificati. *(Applausi del

pertanto l'esame degli emendamenti con altrettanta puntualità e attenzione. L'attività del relatore, anche in Aula, è stata quella di trarre dagli spunti del dibattito elementi per le modifiche normative necessarie, e posso già da ora affermare che l'intenso lavoro svolto tra i colleghi della maggioranza e quelli dell'opposizione porterà a nuove e significative convergenze su alcuni punti, che erano rimasti aperti, che avevo già individuato nella mia relazione iniziale e che altri colleghi avevano rilevato nei loro interventi. È stato questo il lavoro intenso svolto anche in queste ore e in questi giorni per produrre un risultato condiviso. Non mi soffermo, in sede di replica, sulle questioni specifiche che sono state oggetto di ulteriore dibattito e condivisione, limitandomi ad enunciarle. Abbiamo raggiunto un'intesa sulla questione delicata e rilevante del Patto di stabilità,

Non ho altro di sistematico da aggiungere, perché l'ho fatto nel corso della relazione, se non

dell'enunciazione dei problemi, si è concentrato - come a mio avviso è necessario sempre nel lavoro parlamentare - sui testi normativi così da produrre un testo che è il risultato del dibattito e della convergenza delle opinioni. Per questa ragione termino

il Parlamento quand'è stato chiamato a importanti riforme di sistema, come quella che stiamo affrontando, ad onta di quanto talvolta si legge in giro, ha saputo esprimere energie, competenze e passione davvero di grande profondità. È un segnale che forse non emerge all'esterno, ma chi fa il relatore di una legge può testimoniarlo, e io lo faccio con forza.

l'iniziativa parlamentare sia, in una materia di questo genere, particolarmente rilevante e soprattutto lo strumento per poter conseguire risultati concreti e positivi. Mi si consenta di parafrasare Adam Smith relativamente al clima con il quale viene accolto in quest'Aula il disegno di legge in esame. Il preannuncio di una possibile convergenza di tutte le parti politiche verso un voto favorevole al provvedimento non è assolutamente legato alla benevolenza dell'opposizione oppure alla disponibilità della maggioranza, ma credo dipenda esclusivamente da un preciso interesse di tutte le parti politiche

reali che possano costituire le basi, le fondamenta delle decisioni di finanza pubblica. Questo è il principio fondamentale che muove l'articolato e complesso provvedimento che non solo ha l'ambizione di novellare ampiamente la legge n. 468 di trent'anni fa, ma anche di rivedere, in parte, alcuni fondamenti della legge di contabilità del 1923. signor Presidente, credo che questa sia anche l'occasione per affermare un principio che era stato alquanto dimenticato in una gestione consociativa, in una diversa gestione parlamentare, cioè il principio di responsabilità. segue l'andamento della diversa forma di governo che si è affermata negli ultimi vent'anni nel nostro Paese, sancendo con chiarezza la divisione tra la responsabilità delle scelte e della loro attuazione e la responsabilità dei controlli in modo che non vi possano più essere cogestioni nelle decisioni e quindi scarichi di responsabilità con l'unico effettivo risultato - come ha accennato poca fa il collega Baldassarri - di una espansione della spesa pubblica che, in qualche modo, viene posta a carico delle generazioni future. in cui si attua la decisione di spesa e la decisione di bilancio, avere con certezza la contezza degli oneri che essa andrà a comportare, dei suoi effetti sulla fiscalità e sul debito pubblico è assolutamente essenziale per poter dare un ordinato andamento alle nostre decisioni, tanto più in un periodo di difficoltà economica, se non di crisi, come quello attuale nel quale occorre in massimo grado essere cauti relativamente ad ogni possibile espansione della spesa, ad ogni possibile misura che vada ad ostacolare un ordinato fluire dei conti pubblici, perché è chiaro che questo non potrebbe che riflettersi in modo negativo o sull'andamento complessivo del debito, oppure sull'incremento indispensabile del livello di tassazione nel tempo T+1, quando gli effetti di un'eventuale norma espansiva della spesa saranno esauriti. Detto questo, nel ribadire che è di particolare soddisfazione per il Governo constatare che il Parlamento nella sua autonoma decisione è in grado di definire delle norme attuative sulle regole e nel dimostrare, quindi, la permanente validità dello strumento parlamentare anche in un periodo nel quale esso è sotto accusa da parte di molti credo che una legge come questa abbia un significato molto più ampio anche rispetto al suo contingente contenuto), faccio presente che, a mio sommesso avviso, la parte più importante di questo provvedimento è quella in base alla quale si passa da un meccanismo di contabilità di Stato, cioè settore Stato‑Ministeri in senso stretto, ad un sistema di contabilità pubblica. da una parte, a livello di spesa pubblica, la spesa dello Stato è circa la metà del totale intermediato rispetto al PIL (quindi è necessario ricomprendere tutti i soggetti che operano nella pubblica amministrazione e collegarli strettamente), dall'altra, a livello europeo, dobbiamo rispondere in termini di pubblica amministrazione. Pertanto, non avrebbe più senso - e questo è proprio uno dei cardini di questa legge, rispetto al quale un'eventuale modifica significherebbe svuotare assolutamente il contenuto della legge medesima - procedere senza procedere senza una saldatura tra gli obblighi a cui dobbiamo rispondere a livello europeo e i rapporti esistenti tra i diversi livelli di autonomia, vale a dire Stato, Regioni ed enti ed enti locali. La legge consente non certo di decidere che cosa devono spendere le Regioni piuttosto che i Comuni, ma di avere la stessa classificazione dei conti in modo che questi possano essere confrontabili e, soprattutto, si possa sapere effettivamente - e credo che ciò sarà indispensabile anche in fase di attuazione del federalismo fiscale - qual è l'impatto sull'entrata e sulla spesa di ciascun livello di governo. È una misura indispensabile perché,

per centri di costo - che sostanzialmente si guardava l'ombelico ed era costruito sull'amministrazione - ad un bilancio per funzioni rispetto al quale i cittadini possono sapere quanto si spende per questa o quella funzione consentendo

la definizione di conti pubblici più chiari, di una maggiore trasparenza, di una maggiore visibilità, la definizione di organismi di controllo a disposizione del Parlamento tali da consentire a tutte le parti in gioco di confrontarsi a carte scoperte;

anni, oserei dire, è mancata una vera e propria cultura del rendiconto. Il Parlamento e il Governo si accontentavano di votare leggi e il bilancio; poi quello che succedeva succedeva, nessuno si interessava degli effetti. Invece, con il sistema anche l'amministrazione sarà tenuta a comportarsi meglio, perché saprà di essere controllata molto più di prima, perché, certo, è importante decidere come si spenderanno i soldi, ma è soprattutto importante come questi soldi sono stati poi

riportare al centro dell'attenzione il bilancio dello Stato affiancato dal bilancio degli altri enti pubblici in modo da costituire una sorta di consolidato generale del settore della pubblica amministrazione

di definire una sorta di clausola di salvaguardia talché, se nell'applicazione della normativa la spesa eccedesse il preventivato oppure - cosa accaduta molto spesso in passato interventi di carattere giurisprudenziale tendessero ad una espansione della spesa, la suddetta clausola consente di parametrare gli interessi. Fino ad ora molti interventi espansivi della spesa sono derivati da un'applicazione anche in sede di giurisprudenza costituzionale dell'articolo 3 della Costituzione, su cui non

"salvezza" del bilancio vanno contemplate anche nel momento in cui si evidenziano ragioni di eguaglianza che impongono una diversa distribuzione di spese decisa dal Parlamento.

Grazie, dopo trent'anni di continui stress finanziari, anche della sola definizione di legge finanziaria in legge di stabilità, segni in qualche modo una sorta di rappacificazione dei rapporti non solo politici ma anche di approccio rispetto ad una materia che è stata troppo oggetto più di incursioni nei confronti dei *mass-media* e della pubblica opinione che di valutazione concreta degli effetti. Certo, non si può passare da una legge finanziaria a una sorta di legge di serenità, che sarebbe improprio, ma passare ad una legge di stabilità, cioè ridare ai cittadini quella sicurezza, quella stabilità rispetto a un ordinato andamento dei conti pubblici e a un'ordinata gestione, credo sia indispensabile per affermare nel nostro Paese quei princìpi di democrazia economica che fanno sì che solo attraverso la conoscenza dei dati e la condivisione delle regole si possa costruire, ognuno nella diversità dell'opinione, ognuno nella logica diversità degli approcci di politica economica, quel *idem sentire* che alla fine fa il tessuto di una Nazione.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime un parere non ostativo».

Presidente, noi abbiamo presentato più emendamenti per salvaguardare le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Come sappiamo, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno, nelle materie di contabilità e finanza pubblica, competenze particolari regolamentate dai loro Statuti e dalle rispettive norme di attuazione.

Non faremo mancare il numero legale per la ragione che questa riforma, attesa da trent'anni, non è ascrivibile alla maggioranza. Vorrei quindi evitare che su questo si impegnasse anche un pezzetto di campagna elettorale per i ballottaggi che peraltro abbiamo costruito insieme, è ascrivibile alla responsabilità del Senato, maggioranza e opposizione, e il segnale più evidente di questo sta nel fatto che non chiediamo la verifica del numero legale.

4.0.101 (testo 2).

proposta emendativa. La finalità è quella di garantire un più elevato livello di trasparenza delle cosiddette previsioni di consenso che vengono messe alla base delle previsioni sull'andamento dell'economia negli anni futuri.

suo parere contrario.

mi permetterà il senatore Morando una simpaticissima battuta. A conferma che l'unica sua previsione sbagliata nell'intervento di ieri era che non si sarebbe andati indietro, mentre era corretta

che per ora non era mai stato introdotto nella legislazione vigente, in base al quale s'introduce in legge un vincolo per cui il Patto di stabilità interno è derogabile a livello di singolo ente a condizione che il settore nel suo complesso - ad esempio l'insieme dei Comuni, l'insieme delle Province - rispetti il vincolo imposto dal Patto. Si può inserire una forma in base alla quale una quota d'indebitamento dell'ente locale locale viene accollata da uno o da altri enti locali della stessa Regione e, in questo modo, il bilancio complessivo del singolo comparto rimane uguale. Ripeto che si tratta di un principio altamente innovativo, che insieme a tutta la Commissione abbiamo convenuto essere un'ottima novella legislativa in un argomento così delicato come il Patto di stabilità interno, che introduce soprattutto la possibilità di andare a commisurare le diverse esigenze dei diversi enti locali in una condizione attualmente di rigidità complessiva.

In particolare, l'emendamento 9.100 chiede di migliorare ulteriormente il testo per scandire meglio il passaggio tra le previsioni macroeconomiche tendenziali, le previsioni di finanza pubblica tendenziali e le previsioni

della pressione fiscale. Abbiamo constatato che magari si possono vincere le elezioni affermando che si riduce la pressione fiscale, ma

L'emendamento 9.102 intende definire i limiti della pressione fiscale complessiva che sono dati dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il prodotto interno lordo, in modo che esso possa configurarsi sia in termini tendenziali che programmatici, assicurando il rispetto di tale limite. L'emendamento 9.110 va nella stessa direzione, prevedendo una gestione rigorosa dei conti pubblici che riduca la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva: entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa

Abbiamo visto che in un anno il debito pubblico è aumentato di ben 89 miliardi di euro, che equivalgono a quattro manovre finanziarie,

associazioni nazionali dei comuni e si pone un obiettivo molto semplice, partendo da un presupposto chiaro, evidente ed ormai acquisito, e cioè che

su cui, nel corso dei lavori della Commissione e del dibattito in Aula, non siamo riusciti a trovare una convergenza. una convergenza. Presentiamo dunque questo emendamento, insistendo per il voto, ma in un contesto nel quale, ripeto, su questo punto, né con il Governo, né con la maggioranza tramite il relatore, siamo riusciti ad addivenire a un accordo. Per spiegare ai colleghi di cosa si tratta, vorrei sottolineare che il problema non è soltanto quello di introdurre - perché questo problema viene risolto dalla legge e, ad esempio, tanto più dall'emendamento 9.109 del relatore relatore - a fini conoscitivi nella Decisione di finanza pubblica un *target* di pressione fiscale complessiva che non possa essere superato ad orientamento del Governo e della maggioranza, quando quest'ultima avesse approvato quei testi. Il punto che abbiamo sollevato è un altro: riguarda l'introduzione nella Decisione di finanza pubblica e nella conseguente Risoluzione di approvazione della stessa Decisione, per ognuno degli anni di riferimento, un obiettivo di pressione fiscale separatamente dall'obiettivo di spesa, decidendo gli obiettivi per ognuno degli anni in modo vincolante per le entrate e per la spesa.

fosse approvato questo emendamento e fosse introdotto nella legge di contabilità - il doppio vincolo separato per ognuno degli anni di riferimento, a partire dal primo, sulle entrate e sulla spesa, avrebbe come conseguenza l'impossibilità che credo sarebbe un fatto positivo, ecco perché insisto sull'emendamento 9.108 - di presentare durante la sessione di bilancio emendamenti di spesa coperti con aumento di entrata, imporrebbe l'obbligo, qualora in Parlamento si presentassero emendamenti che aumentano la spesa rispetto al tendenziale a legislazione vigente, di coprire quegli emendamenti con corrispondente riduzione di spesa. È del tutto evidente, signor Presidente, che si tratta di una innovazione molto radicale rispetto alla legislazione vigente, alle procedure e alle prassi in corso. Una innovazione che continuo a ritenere necessaria in un contesto nel quale negli anni che ci stanno alle spalle, per responsabilità molto diffuse nei diversi schieramenti politici, abbiamo sistematicamente chiamato le entrate ad inseguire, attraverso l'aumento della pressione fiscale, la spesa che sistematicamente aumentava. Ciò non certo per colpa del Parlamento, che, com'è noto, da quando è stato approvato lo strumento del non realizza nessun assalto alla finanza pubblica, perché mai dal 1978 ad oggi è accaduto che il Parlamento peggiori i saldi della manovra; quindi, non è vero che vi fino ad oggi l'assalto alla diligenza del Parlamento. È vero invece che nel corso della manovra, consentendo di compensare aumenti di spesa con aumenti di entrata, abbiamo spesso fatto lievitare, nel corso della discussione parlamentare, il livello della pressione fiscale. Attraverso questo emendamento noi riorganizziamo la legge di contabilità separando l'individuazione dell'obiettivo di pressione fiscale massima dall'obiettivo di spesa (in particolare di spesa corrente primaria massima), in modo tale che per il futuro si interromperebbe la prassi di far inseguire alla pressione fiscale l'aumento della spesa. Non è che il Governo e la maggioranza non condividano in astratto questo orientamento. Se ho capito bene, nella discussione svoltasi fino ad ora, fino ad ora, lo considerano un mutamento troppo radicale per essere già convenuto in questa sede. Vorrà dire che dovremo fare, spero, per scelta politica ciò che proponiamo qui di fare con l'introduzione di una apposita norma senatore Baldassarri, si tratta di una elaborazione di lungo periodo che viene da lontano nel caso nostro e che non ha avuto bisogno delle sue folgorazioni.

la Decisione di finanza pubblica deve essere approvata dalle Camere: questo è pacifico ed è una questione affidata ai Regolamenti parlamentari.

statale e, infine, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;».

il Governo è d'accordo con la proposta del relatore, pur facendo presente che l'argomento del livello della pressione fiscale, sicuramente fascinoso, comporta effetti pratici non da poco. Ad esempio, in un periodo come l'attuale, nel quale cala il PIL e si modifica il denominatore, è chiaro che saltano tutti i parametri. Per cui il riferimento non può che essere - e non potrebbe essere altrimenti - di carattere indicativo. Non sarebbe infatti un domani, nel momento in cui varia la pressione fiscale in conseguenza della variazione del PIL, restituire delle imposte pagate; sarebbe forse bello per i contribuenti ma sconvolgente sotto il profilo generale. da un punto di vista di principio, un andamento orientato alla diminuzione della pressione fiscale è condivisibile da parte di questo Governo, e credo anche dal Paese, perché ormai è una tendenza che con le difficoltà si cerca di affermare, però praticamente comporta qualche effetto non semplice e facilmente risolvibile.

centrale dell'indicazione di massima della pressione fiscale e della spesa corrente. Questa è la più radicale e profonda modifica della legge n. 468, che si limitava ai saldi. In questo caso introduciamo anche delle indicazioni su pressione fiscale e spesa

da parte del relatore di quell'aggiunta alla lettera *e)* contenuta nell'emendamento 9.100 è positivo dal nostro punto di vista. Tuttavia, vorrei segnalare ai colleghi che

preclusi, restano intatte dal mio punto di vista, malgrado l'approvazione di questa parte dell'emendamento Baldassarri. E ciò

a fini conoscitivi un impegno del Governo nella definizione del livello massimo di pressione fiscale per ognuno degli anni di riferimento, perché comunque, sia pure a fini conoscitivi, rappresenta un elemento di trasparenza nel rapporto tra Governo, Parlamento, cittadini, sistema delle imprese, insomma sistema economico italiano di grande rilievo. Ma la proposta che abbiamo avanzato noi non è di introdurre quell'obiettivo a fini conoscitivi. La proposta che abbiamo avanzato è tesa ad introdurre un obiettivo separato per le entrate e per la spesa che costituisca vincolo alle successive decisioni di bilancio. Quindi è una proposta assolutamente diversa da quella che, pur positiva, in questo momento viene approvata. È chiaro che quindi insistiamo, malgrado quello che è accaduto poco fa, sull'approvazione dell'emendamento 9.108 per le ragioni che ho cercato di spiegare poco fa.

BALDASSARRI *(PdL)*. Signor Presidente, non è del tutto corretto quello che ha detto il collega Morando, nel senso che avendo già incorporato l'indicazione di massima sulla spesa corrente e sulla pressione fiscale la differenza in questo emendamento è che si chiede l'articolazione di pressione fiscale e spesa corrente per singole amministrazioni centrali, locali ed enti previdenziali. Questo *ex ante* è praticamente impossibile. Per questo il mio voto sarà contrario.

e la scansione temporale della presentazione alle Camere di questi documenti nonché la procedura che sotto molti aspetti viene innovata. Pertanto, attribuire un carattere di certezza in termini temporali all'approvazione della Decisione di finanza pubblica nella nuova legge di contabilità sarebbe stato utile. In ogni caso il mio voleva e vuole essere solo un contributo

che tale sia - non ho difficoltà a ritirare l'emendamento

Collega, se lei mi dice di chi si tratta, io intervengo; se non me lo dice, non lo posso sapere, non ho ancora queste virtù divinatorie. A chi si riferisce, collega? Mi dica il nome.

gli enti locali territoriali e per le Regioni. Abbiamo approvato in via definitiva poche settimane fa il provvedimento sul federalismo fiscale e a noi sembra che questo emendamento corrisponda allo spirito di un disegno di legge che abbiamo voluto accompagnare con la nostra astensione e, rispetto al quale, cogliamo gli elementi anche di vitalità di un riordino in senso pluralistico e autonomistico del nostro ordinamento.

il nostro Governo, era allora ministro dell'economia Tremonti, realizzava la più grande operazione di riciclaggio di Stato, facendo rientrare i capitali illeciti frutto di contrabbando con una tassazione del 2,5 Ora rispunta lo scudo fiscale. Il nostro emendamento 14.0.100 ha la finalità di condurre la lotta all'elusione e all'evasione fiscale. Intenderebbe potenziare l'attività del Governo in relazione al contrasto a tali attività e darebbe mandato al Ministro dell'economia e delle finanze, in occasione della presentazione della Decisione quadro di finanza pubblica,

che questo provvedimento si trasformasse più che in una norma esecutiva in una serie di compiti di studio, che poi aggravano il lavoro degli uffici

nel senso che dobbiamo continuamente inserire, quasi come norma di chiusura, la dizione: «fatte salve le prerogative delle Regioni e delle Province a statuto speciale».

L'alternativa è che le Regioni e le Province speciali, di fronte ad un'applicazione errata, ricorrano alla Corte costituzionale per far valere il conflitto di competenza. Non c'è dubbio che le norme attribuite alle alle autonomie speciali derivino dalla forza dei loro Statuti, quindi da leggi costituzionali. Per cui qualsiasi norma ordinaria che questo Parlamento dovesse emanare in contrasto con quelle

sanitario nazionale, ma provvedono con risorse proprie alla gestione e all'organizzazione della sanità. Se in questi ambiti la sanità è completamente regionalizzata o provincializzata, non si capisce perché nel collegio dei sindaci perché nel collegio dei sindaci delle aziende sanitarie o delle aziende ospedaliere debba entrare un rappresentante del Ministero, a rappresentare lo Stato che nulla dà in termini di risorse e di finanza e nulla riceve per l'ambito sanitario. Secondo noi, c'è stato un piccolo refuso. Pertanto, prego il relatore ed il Governo

delle Province autonome di Trento e Bolzano. La seconda è che il riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano non è un'imposizione, è anzi la previsione che esse stesse

parto da quel mistero degli ultimi trent'anni poggiato sull'articolo 81 della Costituzione e sulla legge n. 468 del 1978 che stiamo riformando in termini epocali. si chiede, infatti, come mai con l'articolo 81 della Costituzione, la cui vestale è sempre stata la Commissione bilancio, legge n. 468, che fissava i saldi di finanza pubblica, in trent'anni il debito pubblico in Italia è raddoppiato. Evidentemente, con grande soddisfazione il Popolo della Libertà, il Governo e la sua maggioranza hanno già introdotto il primo pilastro per evitare che accada in futuro quello che è accaduto nel passato. Sto parlando della trasparenza e della chiarezza sull'andamento non solo dei saldi di finanza pubblica, ma anche e soprattutto della pressione fiscale e della spesa corrente. Il secondo pilastro, però, è ciò che viene proposto con l'emendamento aggiuntivo 16.0.100 e cioè una vera e propria Autorità indipendente di certificazione di tutti i bilanci del comparto delle pubbliche amministrazioni, per dare certezza al Parlamento e ai cittadini; e come ho detto in discussione generale questa non è una tecnicalità contabile, ma un pilastro della democrazia e della libertà. Abbiamo pensato andando a realizzare il federalismo fiscale, occorre un'entità indipendente che riferisca al Parlamento e ai cittadini sui bilanci dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti pubblici non territoriali; altrimenti si rischia che quel primo pilastro sulla pressione fiscale e sulla spesa corrente spesa corrente sia parzialmente vanificato dall'incertezza dei dati di bilancio del settore pubblico allargato. Le competenze su questa materia già ci sono; il problema che abbiamo vissuto tutti in questi anni è che le competenze e le responsabilità sulla certificazione dei bilanci sono frammentate, diffuse e in contrasto tra loro; infatti, una parte delle competenze è della Corte dei conti, un'altra è del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, un pezzo importante di competenze alla Ragioneria generale dello Stato, un altro pezzo importante è presso la Banca d'Italia e, ancora, un altro pezzo è presso l'ISTAT. In Italia queste competenze esistono; il problema è che sono frammentate tra loro e non riferiscono in termini unitari al Parlamento e ai cittadini. Si tratta, in realtà, di mettere in coordinamento queste competenze e di dare a questa Autorità la parola certa nei confronti del Parlamento e dei cittadini, che è tutt'altra cosa rispetto a fornire il Parlamento di un adeguato, supportato e rafforzato ufficio studi che coordini, collabori e sostenga l'attività dei parlamentari. Sono due pilastri di una riforma epocale molto importante per il futuro del nostro Paese e, ripeto, sono molto orgoglioso che il mio Governo, il Partito del Popolo della libertà, cui aderisco, abbia avuto la forza, la determinazione e il coraggio di fare dai banchi della maggioranza questo tipo di riforme. Io auspico che si costruisca anche il secondo pilastro di questa riforma che è proposto nell'emendamento 16.0.100: l'Autorità di controllo e di certificazione della finanza pubblica. Non entro nei dettagli dell'emendamento, perché semplicemente articola ciò che ho sinteticamente detto qui pescando le competenze dove già sono, ma unificandole, assegnando ad un'Autorità indipendente il compito di dare numeri certi e impedendo alla politica o al Ministro *pro tempore*, qualunque esso sia, la possibilità di fare quello che ho ricordato in questa Aula poco fa, cioè quello che è avvenuto nel biennio 2006-2007: scoprire tesoretti e sperperarli

link apre una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, per quanto concerne i lavori della prossima settimana, nella seduta antimeridiana di martedì 23 giugno si svolgerà la discussione generale sul bilancio interno e sul rendiconto del Senato. Nella seduta pomeridiana si procederà all'esame degli ordini del giorno sui predetti documenti e alle rispettive votazioni finali. Riprenderà quindi la discussione del disegno di legge di riforma della contabilità e finanza pubblica. **Per lo svolgimento

che si riferisce ai termini e alla relativa applicazione della cosiddetta perenzione amministrativa, esito della legge finanziaria 2008.

proprio ieri il Presidente dell'*Antitrust,* Catricalà, nella sua relazione annuale, ha svolto una severa requisitoria verso un Governo ed una maggioranza che approvano leggi sotto diretta dettatura delle banche, delle assicurazioni e degli altri monopolisti. l'azione di classe doveva entrare in vigore il 1° luglio. È stata rinviata per tre volte e riscritta, introducendo un danno punitivo non, come negli Stati Uniti d'America, verso quelle aziende che frodano il mercato, ma verso i consumatori che osano ricorrere in giudizio. Su questa vicenda abbiamo presentato numerose interrogazioni parlamentari. Se vuole, signor Presidente, cito la

Il rovescio della medaglia, la mancata approvazione dell'entrata in vigore dell'azione collettiva, amplia comportamenti scorretti del sistema bancario: Governo e Parlamento hanno abrogato il pizzo della commissione di massimo scoperto, ciò che i consumatori devono pagare alle banche, surrettiziamente le banche lo hanno reintrodotto, raddoppiandolo di fatto. Allora, signor Presidente, chiedo se per favore volesse la Presidenza invitare il Governo ed i Ministri competenti a venire in Aula per per informarci su quando entrerà in vigore questa azione di classe, che ha già visto tre o quattro rinvii. I furbetti delle banche e dei monopolisti se ne approfittano!

È passato oltre un mese e i due Ministeri sollecitati non hanno dato risposta. Credo che qui dentro qualcuno dovrà ringraziare chi, a partire dalla delegazione radicale, ha imposto

la segretaria dei Radicali italiani Antonella Casu e il segretario dell'Associazione Luca Coscioni Marco Cappato hanno lanciato un appello. Oltre 1.200 docenti italiani lo hanno sottoscritto per chiedere di soprassedere. Se c'è questo movimento di professori (tra l'altro, esiste anche un movimento di studenti fortemente contrario) occorrerebbe avere notizie, possibilmente non il giorno prima la decisione del senato accademico, da parte dei Ministeri competenti in merito alla questione. Sappiamo che si voleva fare un altro regalo al colonnello alla vigilia del G8 della Maddalena. Non si terrà più là. Non si compia nemmeno questa ulteriore possibile vergogna per la Repubblica italiana!

Signor Presidente, vorrei chiedere un interessamento della Presidenza del Senato perché si faccia portavoce nei confronti del Governo, ed in particolare del ministro Sacconi, di una situazione che a Genova sta procurando allarme sta procurando allarme sociale e produrrà una situazione di grave difficoltà. Mi spiego meglio. Da tempo è in atto un accordo di programma, sottoscritto dalla Regione e dal Comune, ma ovviamente anche dal Governo, che riguarda i lavoratori cassaintegrati dell'ILVA.

non sarebbe più concessa a partire da agosto. Stiamo parlando di lavoratori che già oggi mantengono la famiglia con circa 800 euro al mese, quindi con tutte le difficoltà che possiamo immaginare. Non apro una parentesi su chi è catastrofista e chi no e quali sono le situazioni di chi vive la difficoltà

tra l'altro stanno compiendo opere utilissime per il Comune, come lavori ambientali e ristrutturazione delle scuole, quindi stiamo parlando di persone impegnate seriamente anche in lavori molto utili per la collettività),

Signor Presidente, stamattina la stampa nazionale ed anche quella locale (con riferimento ai parlamentari eletti in quelle realtà territoriali)

lealtà che l'attività elencata è riferita solo al dato quantitativo. Malgrado tale premessa, che esonererebbe gli estensori di quel rapporto da qualsiasi giudizio, posto che qualità e quantità non possono essere scissi, anche chi abbia una modesta frequentazione degli ambienti parlamentari, allorché controlla i criteri di attribuzione del voto al singolo parlamentare, si rende conto dell'assoluta inattendibilità, o perlomeno dell'assoluta opinabilità di quei criteri e di quei voti. Basti ad, esempio, precisare che non è dato alcun risalto e valenza, né è presente alcuna valutazione in merito all'attività delle Giunte, che pur sappiamo è un punto di riferimento nodale dell'attività parlamentare.

perché lei in questo momento non vota e quindi, non votando, risulta non solo assente ma addirittura come un parlamentare che non svolge alcuna attività.

sottolineo l'importanza della funzione che dovrebbe svolgere la stampa - neanche la stampa parlamentare, che conosce questi meccanismi e che bene avrebbe potuto valutare i criteri di attribuzione di questa valutazione, ha sentito il bisogno quanto

Senatore Giuliano, lei ha sollevato un tema di particolare rilievo. È ricorrente quest'immagine dell'attività parlamentare

Signor Presidente, avevo chiesto la parola prima che intervenisse il senatore Giuliano per parlare dello stesso argomento, per cui non mi dilungherò. Intendo unirmi pienamente a quanto affermato dal senatore Giuliano e poi da lei, Presidente, sottolineando ancora un altro aspetto di questa inchiesta, ossia quello di mettere agli ultimissimi posti di questa classifica, negli ultimi 20 o 30, colleghi che hanno il 97, il 98 o addirittura il 99 per cento di presenza alle votazioni in Aula, cui vanno ancora aggiunte le cosiddette assenze per missioni, che non sono assenze ma appunto missioni. Si tratta di colleghi che evidentemente, noi lo sappiamo, essendo molto presenti in Aula, sono anche molto presenti nelle Commissioni. Per un verso questa inchiesta sarebbe apprezzabile nell'intento, perché è sempre meglio di ciò a cui assistiamo tutti a cui assistiamo tutti i giorni, cioè del fare di ogni erba un fascio, di dichiarare i parlamentari nel loro insieme, per il solo fatto che sono parlamentari, dei fannulloni, dei mangiapane a tradimento, per usare un'espressione molto elegante rispetto a quello che certi giornali pubblicano. Voglio aggiungere che purtroppo questa è l'unica finestra che viene aperta sui lavori parlamentari, perché per il resto abbiamo una parte del Senato che giace praticamente sempre inutilizzata, ossia le tribune per i giornalisti. Allora ogni tanto forse dovremmo fare una fotografia alle tribune dei giornalisti, che

Certamente i lavori parlamentari si possono seguire anche senza stare nelle tribune, ma le stesse persone che non si degnano di venire a vedere come lavora quantomeno l'Aula (perché ai lavori delle Commissioni solo di rado si può assistere direttamente attraverso le riprese a circuito chiuso) prendono come oro colato quanto viene fatto da tre volenterose associazioni, contro le quali non ho nulla da eccepire perché hanno anche evidenziato i parametri; parametri che evidentemente sono molto difettosi, molto opinabili. Non di meno, mi complimento con i colleghi che sono ai primi posti di questa classifica e io parlo non perché sia stato classificato male, perché anzi sono in una buona posizione in questa opinabilissima classifica. Mi complimento, per esempio, con la collega Poretti che è addirittura al primo posto, che indubbiamente è una parlamentare attiva; però per

stabilito che la presenza non conta niente, l'attività in Commissione non conta niente, presiedere l'Aula, una Commissione o una Giunta non conta niente.

il Comune di Fondi. Da mesi, precisamente dall'ottobre 2008, il prefetto Frattasi ha chiesto lo scioglimento per infiltrazioni mafiose di questo Comune della Provincia di Latina.

e con la *'ndrangheta* di alcuni consiglieri e alcuni addetti amministrativi del Comune di Fondi. Il ministro Maroni, a febbraio, ha accettato la richiesta del prefetto Frattasi per lo scioglimento del Consiglio comunale e l'ha trasmessa al Consiglio dei ministri. Da febbraio 2008 ad oggi non si è mossa più una foglia. Mi dicono che

Tre giorni fa, signor Presidente, l'automobile di un carabiniere che era presente mentre protestavamo è stata fatta esplodere

che ovviamente è ben altro. Però è molto difficile, e soprattutto molto personale, valutare la qualità di un parlamentare rispetto ad un altro. Sui dati e Sui dati e sui parametri utilizzati, fin da ieri si è fatto notare che ovviamente sono migliorabili e gli stessi estensori del rapporto hanno sostenuto che vi erano alcuni vizi; ad esempio ho subito fatto presente che dare un numero così elevato per presentato un disegno di legge ovviamente faceva scendere nella classifica chi ricopre ruoli istituzionali, che solitamente non presenta molti disegni di legge, ed anche i Capigruppo,

che sono disponibili sul sito Internet del Senato, ma non in formato accessibile e quindi prelevabile; quindi non possono essere inseriti in questa sorta di classifica dell'attività dei parlamentari. Tra l'altro,

sono pubbliche, ma ci fu bisogno di parlamentari radicali che mettessero una cornetta davanti alle casse a Montecitorio per mandare via etere e via Radio radicale quello che si discuteva nelle Aule parlamentari. Oggi il

Massimo Cialente vive con 30 dei suoi familiari in uno dei più esclusivi *residence* della costa abruzzese. Il valore del *residence* è di oltre 400.000 euro; il sindaco si è portato con sé 30 persone tra familiari, cugini, fratelli, moglie e associati in un *residence* stupendo. Vogliamo sapere se le dichiarazioni del sindaco rispondono a verità: umiliato forse perché vive in un *residence* stupendo, da mille e una notte, con piscine e idromassaggi, mentre gli altri cittadini sono ancora sotto le tende. Voglio ricordare che il sindaco un paio di giorni è venuto a Roma a manifestare e vorremo sapere se se rientra nella spese della Protezione civile e dello Stato mantenere il terremotato sindaco dell'Aquila con 30 familiari in uno stupendo *residence* con piscine e attrezzature.